sostanzialmente se il Consiglio dei ministri avesse autorizzato l'apposizione del voto di fiducia e su quale testo. una domanda semplice alla quale è stato risposto, peraltro, in maniera non formale dentro quest'Aula dal ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito, che, dopo un'incertezza iniziale, aveva fissato al 25 maggio la data nella quale il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'apposizione del voto di fiducia. Ma la domanda ovviamente non era solo questa: si estendeva, infatti, anche al testo sul quale il voto di fiducia era stato apposto.

del voto di fiducia (strumento ultimo che ha il Governo per ribadire l'assoluta inviolabilità del testo in discussione nell'Aula del Senato, *sub specie* del testo in discussione e del maxiemendamento che il Governo presenta),

questo voto di fiducia viene apposto e rispetto al quale la fiducia stessa è stata autorizzata. Lo dico anche in ragione del fatto che dal 25 maggio ai giorni nostri il testo sulle intercettazioni telefoniche è mutato almeno tre volte e non in forma di dettaglio, tanto è vero che la sua definitiva stesura è stata figlia di una lunga e defatigante discussione all'interno della maggioranza per giungere al testo da sottolineare. Il testo sul quale, non conoscendolo, il 25 maggio il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'apposizione del voto di fiducia è un testo sul quale il Presidente del Consiglio medesimo che chiede la fiducia - o meglio l'ha chiesta, se è vero, il 25 maggio - si è astenuto, come ha avuto modo di dichiarare a tutte le televisioni italiane (e immagino straniere, conoscendo quanto sia proclive rispetto alla comunicazione di massa), insistendo sul fatto che è un testo che lui non condivide, ma che per amore di patria aveva lasciato che l'assemblea politica del Popolo della Libertà approvasse. Questa è una situazione strana. Mi è stato detto dal senatore Quagliariello che io sarei causidica e anche un po' strumentale. Vorrei ricordargli che questione identica o molte volte analoga è stata sollevata da quei banchi anche da autorevolissimi rappresentanti. Ma la mia domanda era molto facilmente solvibile. Sarebbe bastata una nota, proveniente dal segretario del Consiglio dei ministri, come io ho chiesto formalmente in Conferenza dei Capigruppo - in questo caso il sottosegretario Letta - che mi dicesse

Come ho informato ieri l'Aula, ho fatto un riscontro sul comunicato stampa del 25 maggio, ma sul comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 25 maggio non c'è traccia di fiducia. Allora, con i mezzi artigianali che ho a disposizione, sono andata a cercarmi gli altri comunicati stampa del Governo in occasione delle diverse - molte - fiducie che questo Governo ha posto e, in realtà, devo dire che molto correttamente tante e tante volte - questi elementi sono ovviamente a disposizione dei colleghi - il il Governo Berlusconi ha scritto nel comunicato stampa: il Consiglio dei ministri, appositamente convocato, ha deliberato l'assenso a porre la questione di fiducia sul disegno di legge, e così via; questo, più di una volta. Mi potrebbe essere obiettato: sì, è vero, però quando si pone in maniera così preventiva la possibilità di apporre un voto di fiducia, soprattutto perché la maggioranza è recalcitrante e ci sono problemi politici dentro, forse per opportunità è meglio non pubblicarlo sul sito del Governo nel comunicato stampa relativo a quel Consiglio dei ministri. Benissimo, lo capisco, ma allora, con molta grazia istituzionale, sarebbe potuto accadere ciò che io ho chiesto, e ho chiesto anche in maniera molto cortese, educata, rispettosa delle regole istituzionali. Presidente, Presidente, non vorrei metterla in imbarazzo: quando lei era Ministro per i rapporti con il Parlamento e il collega Malan aveva sollevato analoga questione, gli arrivò tempestivamente, a stretto giro, una nota

che in tale data, effettivamente era avvenuto. Una sorta di estratto del verbale del Consiglio dei ministri, perché così si ragiona nella civiltà delle relazioni istituzionali, invece, ora non è accaduto. Io non sono stata destinataria né di una missiva e neanche di una telefonata di cortesia. Il presidente Schifani è stato ovviamente tenuto fuori da tutta questa *bagarre*; ha sottolineato più volte, il presidente Schifani, un atto rientrante fra gli *interna corporis* e che, quindi, il Presidente non ha nessuna responsabilità. Devo dire, per memoria storica, che nella scorsa legislatura

di sollecitazioni che noi evidentemente ci permettiamo di anticiparle - sotto il profilo del controllo della legittimità del percorso, l'effettiva sussistenza di un'anomalia procedimentale, ritengo che andrebbe addebitata non tanto una responsabilità politica al Governo quanto una responsabilità endoprocedimentale alla Presidenza del Senato, trattandosi di una legge che esce da questo ramo del Parlamento». In un intervento colto e motivato,

Ma - ripeto - tutto questo avrebbe potuto essere pienamente risolto con una missiva di poche righe proveniente dalla Presidenza del Consiglio; invece non l'abbiamo ricevuta. A questo punto avanzo un'altra domanda. Per quale motivo non l'abbiamo ricevuta? Perché così come si tiene «in gran dispitto» la Costituzione, si tiene «in gran dispitto» anche il Parlamento e il Capogruppo del maggior Gruppo dell'opposizione che pone una questione seria.

la legge n. 400). E se deve spostare l'oggetto della fiducia o mutare l'atteggiamento del Governo rispetto al testo, ha bisogno di essere nuovamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, che peraltro è in corso, e quindi avremmo potuto fare a meno di tanta sgradevolezza, se soltanto avessimo voluto. Da ultimo, Presidente, siccome ci tocca

Questo precedente della Giunta del Senato lo trovo particolarmente interessante perché incide esattamente sulla questione sulla quale stiamo ragionando. Ne leggo solo poche righe: «La questione di fiducia non instaura un dibattito a sé stante, ma diventa la cornice della discussione

tra la conoscenza, quell'oggetto e il voto. «La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenzaۛ (...)». Credo di aver

le chiedo di investire anche il Presidente del Senato della convocazione della Giunta per il Regolamento, per dipanare una questione che, tra troppi equivoci e troppi lassismi, rischia di trasformare una cosa seria in una farsa.

I procedimenti che riguardano l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo appartengono, come si dice in dottrina, agli *interna corporis* del Governo. In sostanza, la questione riguarda il Consiglio dei ministri. Il Ministro che rappresenta il Governo in Parlamento pone la questione di fiducia - può farlo il Presidente del Consiglio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento (questo è l'uso), talvolta anche lo stesso Ministro di settore - e, dal punto di vista della

in un altro in quella sede, perché a quel punto si intende che comunque il Governo nella sua collegialità ha delegato il Ministro competente - in questo caso il Ministro per i rapporti con il Parlamento - a porre la fiducia e, non essendo smentita, questa

un atto della Presidenza del Consiglio che venisse trasmesso alla Presidenza del Senato in cui si dicesse, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che attesta i verbali del Consiglio dei ministri, che effettivamente in quella data è stata richiesta, e ne è stato dato mandato al Ministro competente, di porre la fiducia. Questo è il punto che ci riguarda come procedura. La Presidenza del Senato ha chiesto all'ufficio del Ministro per i rapporti con il Parlamento il verbale,

Signor Presidente, non voglio aggiungere altro a quanto ha già detto il Presidente del nostro Gruppo, vorrei solo sottolineare il disagio di chi si è sottoposto ad una serie di sedute inutili della Commissione giustizia quando già, a quel che si apprende, la fiducia era stata autorizzata ad essere posta dal 25 maggio del 2010. Credo sia un atto gravissimo nei confronti della dignità del Parlamento ed in particolare dei componenti della Commissione giustizia, che sono stati sottoposti ad un lavoro assolutamente inutile per ben tre sedute, con rinvio del provvedimento dall'Aula in Commissione senza alcun beneficio per il testo, se non la risoluzione dei problemi interni della maggioranza che evidentemente aveva gravi difficoltà a trovare, come si dice, la quadra. Tre sono i profili che il nostro Gruppo ha sempre posto all'attenzione dell'opinione pubblica.

fatti della vita privata dell'indagato o di terzi, potessero entrare a far parte di atti di indagine ed essere poi improvvidamente pubblicati.

illegali, garantire la libertà di informazione intesa da una parte come diritto di informazione garantito costituzionalmente per la stampa ma al contempo, come diritto dei cittadini ad essere informati di quanto effettivamente accade nel Paese e in particolare del malaffare. Tutti questi valori sono costituzionalmente garantiti, in particolare il diritto da parte del cittadino valutare l'attività dell'organo giurisdizionale, di fare quel controllo sulla giurisdizione che gli spetta, perché in nome del popolo italiano viene amministrata la giustizia, di fare nel contempo il controllo sulla cosa pubblica che gli deriva dall'essere quel popolo sovrano che nomina i propri rappresentanti politici rispetto ai quali ha diritto di ottenere risposte coerenti con il mandato che viene conferito e, soprattutto, di mutare opinione politica quando questo mandato viene tradito. Ha diritto, altresì, di controllare ciò che la cosa pubblica fa e quindi ad una trasparenza e correttezza dell'attività della cosa pubblica, che è un altro valore costituzionalmente garantito.

all'unanimità alla Camera e poi approfondito in Senato e che decadde solo per la fine della legislatura stessa) e ai disegni di legge presentati in questa legislatura, uno da me con il senatore Ceccanti, che riprendeva i principi del disegno di legge Mastella con aggiornamenti alla luce del dibattito parlamentare che c'era stato;

Il disegno di legge che vi accingete ad approvare, che è costituito da un maxiemendamento che sostanzialmente ripropone il testo della Camera con qualche piccola modifica, non risponde ad alcuno di questi requisiti.

Tutto ciò contrasta naturalmente con un principio di ragionevolezza anche rispetto alla conclamata volontà di avere tempi rapidi nell'esercizio della giurisdizione, di garantire una giustizia rapida oltre che agli stessi imputati che hanno diritto anch'essi ad un giusto processo e che possono essere trascinati, da coimputati, in vicende che nemmeno li riguardano, ma che sono

vuole liberarsene, cercando di rallentare il corso del processo e giovarsi così della prescrizione, e il gioco è fatto. Consentendo tutto questo, naturalmente, il processo si rallenta, il diritto alla sicurezza dei cittadini viene posto in seria discussione

non c'è nessuna violazione del segreto di indagine e non c'è neppure, da parte dei giornalisti che li pubblicano, un reato di arbitraria pubblicazione.

non si comprende per quale motivo, se si tratta di atti conosciuti ai difensori e agli indagati, essi non possano essere oggetto di discussione pubblica e quindi anche di valutazione della pubblica opinione attraverso le informazioni pubblicate dagli organi di stampa.

e atto pubblico: si viene a creare una sorta di limbo, in cui atti che non sono più coperti da segreto e che sono anche assolutamente pertinenti alle indagini e ai reati

quel sistema di rapporti impropri tra magistrati, cancellieri, giornalisti, avvocati, personale giudiziario, collaboratori degli avvocati che dà vita a quella deprecabile compravendita della notizia

giustizia senza nessun vantaggio per la sicurezza dei cittadini, che viene indebolita, per la *privacy* di coloro che vengono chiamati in causa e per la libertà

è antidemocratico e non può essere accettato da un Paese civile. non ripercorrerò i punti salienti di questo provvedimento, che sono stati sviscerati anche adesso e in tutto il corso del dibattito pubblico e nelle Commissioni (non tanto in Aula, in cui siamo arrivati in questo modo). Mi consentirete, però, colleghi, qualche commento politico di ordine più generale. Siamo arrivati quindi al punto finale, ampiamente annunciato, con l'apposizione della questione di fiducia, ammesso sempre che arrivi il fax. Anzi, signor Presidente, quando arriva la comunicazione via fax

So bene di utilizzare una parola molto pesante, ma, colleghi, la procedura e il metodo con cui siamo arrivati ad oggi non esito a definirli demenziali

che qualcuno formalmente dichiari che la questione di fiducia è stata posta il giorno X sul testo Y. Neanche questo riusciamo a sapere. Dopo il delirio, il guazzabuglio di emendamenti presentati, ritirati, modificati, modificati, molto spesso assurdi, irrazionali, siamo arrivati a questo giorno e a questo voto. Il metodo, quindi, è ben lungi dell'essere un minimo aderente a quello che in un Paese normale viene definito un dibattito democratico, in cui ci si scontra su posizioni diverse, ma si è legati sulle regole

È una fiducia posta perché non ve la sentivate di affrontare voti segreti. È una fiducia posta perché non è consolante per nessuno, anzi desolante perfino per voi, sapere che dietro c'è stato, forse ieri, un accordo. Patti, accordi, tregue, punti di equilibrio: sempre dietro, perché davanti questo testo punti di equilibrio, di razionalità e di aderenza costituzionale non ne presenta di sicuro. L'imbarazzo vostro è tale avete dovuto - qui e probabilmente anche alla Camera - chiudere a qualunque tipo di obiezione puntuale da parte di vostri colleghi della maggioranza su un testo inaccettabile. Inaccettabile per molti di voi, oltre che per noi. Questo è un altro segno di una china rovinosa, che mi pare stia accelerando ogni giorno, in cui sempre di più sembrate scambiare la forza dei numeri con il diritto.

non devo commentare: l'arroganza con la legalità. Il testo tende anche a scambiare la libertà individuale con la licenza

che questo è un provvedimento teso semplicemente all'oscuramento che avete perfino inserito norme che con le intercettazioni telefoniche non c'entrano nulla. Mi riferisco alla nota questione della registrazione dei processi: onorevoli colleghi, ma a che fine, se non a quello dell'oscuramento? La prassi attuale da noi praticata da anni non ha dato mai - mai - esito a contestazioni. il dibattimento processuale è pubblico, dice la Costituzione. Che bisogno c'era di oscurare, se non per questa idea di fondo per cui l'oscuramento deve guidare l'esercizio della politica in questo Paese?

E non si capisce neanche l'obiettivo di tutto questo, se non questa pervicacia, questa crisi rovinosa (secondo me, ormai), questa china rovinosa che sembra non avere più limiti. ammesso che il voto che vi apprestate e ci apprestiamo a dare abbia presupposti di legittimità e di legalità, in attesa del noto chiarimento,

più, sono convinta che questo provvedimento, nell'ulteriore passaggio alla Camera, richiederà altri equilibri, come si dice, altri punti di accordo. Tutto ovviamente in modo extraparlamentare, perché qui siete sopratutto chiamati a ratificare, a ratificare per esempio, persino un Presidente del Consiglio che non si riconosce nel testo, tanto è vero che non lo approva e dichiara *urbi et orbi* che non lo approva e non è il suo testo; dopo di che, povero, senza potere com'é, com'è evidente, pone la fiducia. E questa Camera che deve fare, secondo voi? Ma che dobbiamo fare semplicemente per richiamarvi ad un minimo di decoro istituzionale che dovrebbe essere nel patrimonio di tutti, destra o sinistra che sia? Questa è la china rovinosa che oggi, di giorno in giorno, di volta in volta accelera. Capisco il vostro disagio. Capisco quindi che, in violazione della Costituzione, questa fiducia non è stata posta per i motivi che la Costituzione prevede,

che questo è un momento di una lotta che non finisce qui, non solo perché avrà punti di ricaduta nell'altro ramo del Parlamento, ma perché riteniamo, anche da Radicali, che nel Paese debba nascere e crescere una rivolta democratica, una rivolta legale a questa china rovinosa.

la diminuzione del livello di sicurezza nel Paese, il bavaglio che viene imposto alla stampa e la non tutela della *privacy* delle persone. Il primo aspetto è quello che concerne la sicurezza.

perché queste norme incidono ampiamente e in negativo in materia di sicurezza e in materia di lotta alla criminalità. E questo ce lo dicono tutti gli operatori della sicurezza, ce lo ricordano tutti i sindacati di Polizia. Mi limito a ricordare alcuni di questi aspetti. Innanzitutto, ricordo la limitazione delle intercettazioni ambientali in luoghi pubblici, e non per acquisire prove sui reati commessi, ma per quelli eventuali e futuri, quasi ancora *in mente dei*. la limitazione nell'accesso ai tabulati telefonici e la ridicola commedia delle proroghe da richiedere ogni 48 o 72 ore, con i poliziotti e i carabinieri che dovrebbero scorrazzare - con le macchine che magari non hanno, con la benzina che magari non hanno, con il personale che non basta mai - dalla montagna alla periferia di ogni regione fino al capoluogo per richiedere proroghe, con faldoni e faldoni di carte processuali, invece di badare alla prevenzione del crimine e alla sicurezza dei cittadini. Altra limitazione è l'imposizione del tribunale collegiale come giudice competente in materia di intercettazioni, che comporterà disfunzioni, disorganizzazione e rischio di blocco di una macchina giudiziaria già asfittica e impotente. ancora, le limitazioni imposte alla possibilità di intercettare persone non indagate, per così dire quasi indiziate di collegamento diretto con le indagini, e soprattutto le limitazioni imposte con questo disegno di legge alle intercettazioni dei cosiddetti reati satellite o reati spia, fondamentali per arrivare ad accertare i reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Tra questi ricordiamo il delitto di usura, di estorsione, di corruzione: insomma, sostanzialmente i reati della cricca. Prima di passare all'aspetto che concerne la libertà di stampa, voglio soltanto citare un'altra norma pericolosa: quella che consente a qualsiasi indagato, a qualsiasi criminale o terrorista, di eliminare un magistrato inquirente o giudicante scomodo, non gradito, e che consente di far saltare le indagini più complesse, più pericolose per il potere, per i criminali e per i terroristi. Questa norma che voi volete approvare è un'arma concessa ai criminali che rischierà, tra l'altro, anche di condurre a scarcerazioni indebite e pericolose. Il secondo aspetto fondamentale, come dicevo, è quello che concerne la libertà di stampa, il bavaglio che volete mettere alla libera stampa. Mi basti ricordare che sotto dettatura del vostro Presidente del Consiglio - mi verrebbe da dire sotto dittatura del vostro principe state approvando norme liberticide, norme che sono estremamente limitative della libertà dei giornalisti di scrivere e di informare, norme estremamente limitative del diritto dei cittadini di sapere cosa avviene nei palazzi della politica e nei palazzi di giustizia, come norme di trasparenza imposte dalla Costituzione vorrebbero. In particolare, infischiandovene di ogni nostro emendamento, confermate il carcere per i giornalisti e aggravate, con il maxiemendamento finale, le sanzioni per gli editori, in modo palese non solo la Costituzione italiana, ma altresì - e sempre in modo palese - la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il Trattato di Nizza. Ricordo poi che la ormai costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, in sentenze recenti, a partire dal giugno 2007 fino al 2009, sancito che il diritto di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati hanno un rango e un rilievo superiori allo stesso segreto istruttorio quando si tratti di fatti di eccezionale rilievo sociale e politico. La stampa, dice la Corte di Strasburgo, è come *le chien de garde*, il cane da guardia di ogni democrazia. Voi, cercando di eliminare la libertà di stampa e il controllo istituzionale della magistratura, state minando le basi stesse del nostro sistema democratico. Per fare ciò - e vengo al terzo aspetto fondamentale di questo disegno di legge - vi nascondete dietro il falso proposito di tutelare la riservatezza delle persone. Dico falso proposito perché, se davvero aveste voluto tutelare la *privacy*, sarebbe stato sufficiente accogliere almeno i nostri principali emendamenti in questa materia, emendamenti che prevedevano e prevedono, ad esempio, una serie di filtri (almeno cinque) per impedire la fuoriuscita di notizie concernenti fatti o persone estranee al procedimento penale. Inoltre, prevediamo nei nostri emendamenti e nei nostri disegni di legge, come Partito Democratico, tutta una serie di responsabilità che vengono precisate e tutta una serie di sanzioni per le varie fasi delle operazioni delle intercettazioni e per i vari soggetti operanti, magistrati compresi. Ma a voi, in realtà e molto concretamente, non interessava e non interessa tutelare la riservatezza delle persone normali: a voi interessava e interessa tutelare la cricca, i criminali degli appalti, gli affaristi della politica, e per fare ciò fornite un concreto aiuto ai criminali veri e mettete le manette alla polizia, rischiate di far saltare completamente le già derelitte strutture giudiziarie, cercate di bloccare le indagini per voi più scomode e scottanti, mettete un bavaglio alla libera stampa, impedite l'informazione ai cittadini di questa nostra Repubblica. La prova della vostra malafede - perché lo fate dolosamente, tutto ciò - sta nella norma sul regime transitorio che avete introdotto qui al Senato e che avete ribadito con il maxiemendamento. Il regime transitorio è la prova di tutta la fretta che voi avete nel coprire le vostre malefatte, le malefatte della vostra cricca.

«Confermo che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 25 maggio scorso, ha manifestato il proprio assenso a ricorrere allo strumento regolamentare della fiducia, qualora risultasse necessario, in ordine al disegno di legge sulla nuova disciplina delle intercettazioni giudiziarie». è firmata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quindi, dal punto di vista della procedura, è la conferma che il Consiglio dei ministri ha dato questa autorizzazione. Le questioni politiche

Signor Presidente, onorevoli senatori, appartengo, come è noto, a quella esigua e tenace minoranza che cerca di interessarsi del merito dei problemi e non degli strumentalismi che vi fioriscono intorno. la mia sensazione, personalissima, ma credo condivisa da nove cittadini su dieci che eventualmente abbiano seguito tutta questa vicenda, è che alle forze politiche sia interessato più ciò che c'era dietro, o sopra o sotto, che non il merito del provvedimento. Ecco perché (in pochi attimi non posso fare che degli accenni - perché no? - anche polemici) le opposizioni, che ho avuto modo di ascoltare attentamente durante questi mesi di lavoro, si sono divise, sì, in falchi e colombe, ma non soltanto: anche in molti altri tipi di uccelli, onorevoli senatori. I falchi, certo: coloro che nel PD o altrove volevano occupare l'Aula, fare manifestazioni di protesta clamorose. Le colombe: coloro che, più aderenti alle regole e al buon tono, avrebbero voluto fare dell'ostruzionismo corretto, più morbido, più levigato. Ma anche altri tipi di uccelli politici. Certamente vi sono anche i corvi, non sia offesa per nessuno, coloro che giocano al tanto peggio tanto meglio e che sono interessati più che altro a far risuonare qui, per quanto possibile, le voci non del popolo tricolore (magari!), ma del popolo viola, sempre più isterico e disperato, dei "santorini", dei "travaglioidi". Ma ci sono anche altri uccelli: le cinciallegre, quelle che in qualche modo hanno voluto usignolare anche con la maggioranza e con il Governo, ma senza trarne le conseguenze, disposti ad esaminare i testi purché fosse chiaro che restavano comunque su una linea di opposizione.

perché naturalmente è diventata un'arte sofistica anche quella di essere nidi dei cuculi e al tempo stesso riportare a casa - come si suol dire ormai in gergo - i risultati politici di certi dissensi dosati e calibrati.

*(PdL)*. Voterò la fiducia al Governo che, in sintesi, sta assicurando, nonostante le eccezionali difficoltà, la rotta della coesione sociale e del mantenimento degli equilibri economico-finanziari. Ma voterò anche la fiducia al provvedimento, che non è il massimo dei miei sogni personali e dei miei desideri, ma - come dissi ormai quasi un anno fa in Commissione giustizia del Senato - quando si è di fronte agli abusi, agli eccessi e al ludibrio è inevitabile e ci si assume la responsabilità delle reazioni e dei giri di vite che si è necessitati ad adottare. Qualche illustre collega ha sottolineato che con questo provvedimento abbiamo tamponato gli effetti più che curato le cause di certe degenerazioni. Lo so, è la verità! Senza voler insegnare all'opposizione a fare l'opposizione, che è un mestiere che ho svolto per qualche decennio, voglio evidenziare che se l'opposizione avesse inteso

Gli eccessi sono dunque la causa delle reazioni, anche sul piano legislativo. Voto il provvedimento perché esso argina gli abusi incontenibili che si sono verificati, oltre alla dilapidazione di risorse o comunque al dilagare di una voce di spesa che ormai è diventata la prima di un bilancio della giustizia sul quale pure spesso versiamo lacrime e facciamo proteste fondate. perseguire indagando, tornando ad indagare, e non affidandosi soltanto alla generica rete a strascico delle intercettazioni. tutelare il bene della riservatezza e della privatezza, che è proprio delle società libere (è inutile fare ossequio a parole a questo principio e poi sottostimarlo) contro lo scempio che se ne fa quotidianamente anche da parte - perché no? - di mezzi di informazione che dovrebbero essere rigorosi con loro stessi ed essere strumenti di informazione e di crescita democratica e non di aggressione ai singoli e Si deve agire contro i traditori del segreto d'ufficio, che è uno dei più gravi delitti, carissimi colleghi, che può essere commesso da chi vuole onorare certe funzioni che è chiamato a compiere. Mi meraviglia che i molti richiami etici sollevati non si siano soffermati su questo aspetto: il tradimento del segreto sacro del proprio ufficio è uno dei delitti più gravi che si possono registrare in una società moderna, evoluta e democratica. Peccato, dunque, che un ostruzionismo assolutamente puerile abbia condotto a quella che chiamiamo in gergo parlamentare la blindatura del testo finale.

quello che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal competente giudice delle indagini preliminari al tribunale in forma collegiale del capoluogo del distretto. È un errore tecnico evidente, che rischierà di inceppare la legge e di mettere in crisi il sistema, paralizzare taluni tribunali, creare diseguaglianza di poteri tra tribunali, creare traffico e violazioni alla riservatezza. Lo dico con tutta franchezza e non è stato possibile rimediarvi. Ebbene, proprio

Proprio in questi giorni l'Associazione nazionale magistrati, nel criticare questo provvedimento e altri aspetti attinenti alla manovra, ha chiesto di sopprimere i tribunali periferici, di accorpare i piccoli tribunali, di chiudere le sezioni distaccate di tribunale, di chiudere metà degli uffici del giudice di pace

di subire un taglio alle proprie retribuzioni, non per risolvere problemi finanziari ma per dare un segno e un esempio, è veramente ridicolo - lo dico senza demagogie, cari colleghi cari colleghi - che le grida più alte vengano da ceti estremamente sofferenti come gli alti magistrati o i farmacisti urbani. Ci manca soltanto che insieme a voi, campioni del popolo che non arriva alla fine del mese, occupino i banchi del Governo ceti sofferenti come i divi del pallone, i divi della televisione o magari i colleghi del notariato! Allora sì che Di Pietro e Bersani sarebbero veramente i campioni del popolo, schierandosi a fianco di queste grida di dolore! Il cittadino ci inchioda a queste responsabilità e quando si vara una legge dopo molti anni di dibattito, dopo due anni di legislatura e dopo che ci si è confrontati con inutili ostruzionismi,

Queste sono le ragioni (in pochissimi minuti non posso dire di più, ma sono pronto a qualsiasi dibattito e in ogni sede) per le quali si impone, per motivi di merito e di quadro politico, di conferire, formalismo o non formalismo, il voto di fiducia al nostro Governo.

posta dal Governo. In considerazione dell'orario già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo per le dichiarazioni di voto con trasmissione in diretta televisiva, sospendo la seduta fino alle ore 11,30. *(La seduta, sospesa

colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Prima di passare alle dichiarazioni di voto, riscontro che nei banchi del Governo sono seduti molti esponenti di un Gruppo

Invito per la seconda volta i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo a lasciare quei banchi e prendere posto nelle loro allocazioni istituzionali, e li richiamo nuovamente all'ordine. Richiamo nuovamente all'ordine, per la terza volta, i senatori che occupano indebitamente i banchi del Governo e li invito a lasciarli immediatamente, per la terza ed ultima volta. La Presidenza, a questo punto, è costretta

Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, due diritti, entrambi fondamentali per una società civile evoluta, quello alla *privacy* e quello ad essere informati, sono diventati, loro malgrado, antitetici: tesi ed antitesi. Il loro bilanciamento, un bilanciamento adeguato, era quindi necessario e non più rinviabile. Purtroppo i diversi interventi legislativi - penso al codice della *privacy*, ovvero al decreto legislativo del 30 giugno 2003, 196, alla legge del 20 novembre 2006, n. 281, sulle intercettazioni acquisite in modo illegale, agli articoli 114, 115, 329 ed altri del codice di procedura penale, ed anche alla Costituzione con l'articolo 15 - non sono riusciti a comporre gli interessi, che ormai possiamo definire voyeuristici, che, ben oltre il contenuto, si basano ormai sulla mera notizia. Sono anni, onorevoli colleghi, che i magistrati e i giornalisti si palleggiano le responsabilità sulla fuga di notizie, incuranti del fatto che spesso a pagarne le conseguenze è il cittadino, che in molti casi non sarà nemmeno indagato e che, fortuitamente o meno, ha relazioni di qualsiasi genere con la persona intercettata. Così, la storia giornalistica italiana si è colorata di Tangentopoli, Calciopoli, Vallettopoli ed oggi già si parla di una seconda serie rispetto alla precedente indagine per gli eventuali nuovi sviluppi e via via andando avanti. I dati forniti da Eurispes sono impietosi. Vi è un incremento vertiginoso delle intercettazioni

La spesa complessiva nel periodo 2001-2007 è stata di oltre 1 miliardo e mezzo di euro e solo nel 2007 ha raggiunto una cifra pari a poco meno del 3 per cento del bilancio del Ministero della giustizia: circa 225 milioni L'analisi del dato puramente economico non è secondaria ed ha sicuramente un grande effetto sull'opinione pubblica, soprattutto su quella maggioranza di cittadini perbene che non sarà mai intercettata. É anche corretto però sottolineare come questo mezzo sia utile e addirittura insostituibile in molti casi. Dovrebbe emergere forse con più forza e più chiaramente che le spese sostenute per le singole inchieste spesso vengono non solo compensate dal denaro recuperato, ma a volte anche ampiamente superate. Al di là di questi aspetti meramente economici, le intercettazioni restano uno strumento essenziale e la letteratura giuridica, ma soprattutto processuale, può dimostrarne l'importanza, in particolar modo riguardo alla lotta ai reati mafiosi. A tal proposito, l'audizione in Commissione del procuratore nazionale antimafia Grasso aveva dato spunti migliorativi fondamentali per il testo, che noi del Movimento per le Autonomie abbiamo raccolto e presentato sotto forma di emendamenti. Il Governo ha però ritenuto di riassorbirne solo uno nel proprio testo. La maggioranza ha perso un'opportunità, a mio parere, quella non solo di rendere il testo più equilibrato, ma soprattutto di evitare il rischio di appannare i risultati ottenuti in questi due anni di lotta contro la mafia. È mancato il confronto necessario e anche il coraggio di guardare oltre la siepe dei reati satelliti, che così come disciplinati rischiano di limitare e lasciare monchi gli strumenti ad oggi previsti per il contrasto alla criminalità organizzata. Chi come me vive nel Mezzogiorno conosce bene questa piaga,

Questo testo avrebbe dovuto realizzare un compiuto equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all'informazione. Questi diritti non sono stati pienamente raggiunti e proviamo disagio di fronte alla richiesta di fiducia, che esula il contraddittorio necessario su un tema così importante....

ma insufficiente, nell'esprimere disagio e rammarico per l'opportunità non completamente raccolta, il Movimento per le Autonomie non parteciperà al voto. Signor Presidente, intervengo con un po' di imbarazzo rispetto all'episodio di poco fa, perché, per quanto mi riguarda, la democrazia si nutre anche di simboli e, sempre a mio avviso, le Aule parlamentari hanno un significato quasi sacrale per la nostra Repubblica. Quindi, non condivido quello che è accaduto.

Tratta di argomenti per cui bisogna necessariamente ricercare sempre una condivisione più ampia, e non la solitudine con la quale l'attuale maggioranza di forza si appresta ad approvare queste norme. Se il Governo esaminasse quello che accade, senatore Centaro, vedrebbe che nessuna forza politica potrà votare il vostro provvedimento,

con più prudenza, con più ponderatezza. Non è un caso se all'inizio di questa legislatura abbiamo presentato una proposta, che è agli atti del Parlamento, per istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni. proprio perché si potessero trovare, nell'esame di quello che era accaduto, convergenze significative. Il provvedimento oggi al nostro esame riguarda la natura della democrazia nel nostro Paese: per questo è sbagliato approvarlo a colpi di maggioranza o di fiducia, come vi apprestate a fare. Nel merito, noi avremmo votato contro tutte le parti del provvedimento che prevedono limitazioni allo strumento investigativo. Non si può fare a meno di questo strumento o limitarlo, non si può arretrare nella lotta alla criminalità o nella lotta alla corruzione. Avremmo, quindi, valutato caso per caso, emendamento per emendamento, comma per comma, tutti i passaggi di quell'unico articolo, tutte le norme a tutela della *privacy*,riferendoci anche a quanto era accaduto nella scorsa legislatura, a quel provvedimento che era stato presentato dal Governo Prodi e che aveva trovato in un ramo del Parlamento un'ampia, amplissima convergenza.

siamo consapevoli che gli anticorpi, che pure esistono nella magistratura, perché spesso il giudice terzo annulla ciò che succede in alcune procure, persino quegli anticorpi che comunque dobbiamo sempre tutelare, spesso arrivavano tardi, a danno già avvenuto. Siamo persino consapevoli che non riguarda tanto gli innocenti, i terzi che finiscono nelle indagini. E siamo consapevoli che non c'è nessuno

colpevolizzare oltre ciò che prevede il codice chiunque, guardando ai suoi orientamenti, alle sue opinioni, parla di vicende che nulla hanno a che fare con gli episodi per cui si indaga.

Signor Presidente, dietro all'ipocrita richiamo al rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni si demolisce oggi uno dei più importanti mezzi di ricerca della prova dei crimini. La tutela del principio costituzionale andava assicurata con i giusti presìdi in ordine alla riservatezza delle captazioni, con il loro uso ponderato selezionato nel contraddittorio delle parti, con le inasprite sanzioni per le violazioni della segretezza. Il Governo e la maggioranza hanno voluto invece altro e su questo altro non potranno rispondere con onestà alle domande degli italiani. Il Governo si gonfia il petto per gli arresti operati dalle forze dell'ordine - che noi ringraziamo sempre - e dalla magistratura. Ne fa un proprio merito. Ma ora demolisce le norme che quegli arresti hanno facilitato e, spesso, esclusivamente determinato. Vi pongo io le domande che i cittadini vorrebbero farvi e alle quali non potrete rispondere se non con l'inganno. Perché avete reso così difficile, tortuoso e insidioso il percorso per cercare la prova dei crimini? Perché avete, di fatto, cancellato la possibilità delle intercettazioni ambientali, prescrivendo che esse potranno effettuarsi nei luoghi privati solo se vi è il sospetto di attività criminosa in atto, anche se si cercano le prove in ordine ad un delitto già consumato? Perché volete consentire le intercettazioni ambientali solo per tre giorni, sia pure prorogabili, e solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico? Perché non potrà più tentarsi di captare le conversazioni dei sospettati di gravi crimini collocando, ad esempio, la cosiddetta cimice in un'autovettura o in una masseria o in un capannone o in un circolo privato? Perché avete abrogato l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, la cosiddetta legge Falcone, che accomunava, ai fini della possibilità, della durata e delle modalità delle intercettazioni, tutti i fatti di criminalità organizzata, mafiosa e non? Perché avete, con la detta abrogazione, escluso grandi e pericolosi crimini dalla possibilità di intercettazione cosiddetta semplificata? Perché avete voluto annullare una legge di estrema importanza nella lotta al crimine e che l'Italia deve alla felice intuizione di Giovanni Falcone? Perché non avete voluto prevedere l'arresto in flagranza obbligatorio per il reato di pedofilia? Perché prima avete accettato questa norma e poi l'avete cancellata, con la motivazione di ingiusta previsione dell'arresto nei casi di minore gravità e, però, cancellando anche l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i casi gravi di pedofilia? Perché avete voluto reintrodurre in Italia la censura, vietando la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto? Perché non volete che i cittadini sappiano? Perché volete l'omertà di Stato? Perché odiate la libera informazione? Voi non avete una risposta a nessuna di queste domande. Io tenterò di darvi la risposta: perché lo vuole Silvio Berlusconi ed il suo sistema; il protettore adottato dal malaffare; l'uomo che ieri ha detto: «Non c'è stata alcuna cricca, niente di meno che positivo». Ovviamente per lui. Proprio oggi i giornali parlano dell'indagine che riguarda Verdini. L'uomo che ha detto ieri: «Governare con le regole che impone la Costituzione è un inferno». Ho cercato di attualizzare in maniera più sincera una lettura delle dichiarazioni rese ieri dal presidente Berlusconi e ho fatto qualche minimo ritocco: disegno di legge - «in questa direzione perché il diritto alla riservatezza e all'inviolabilità» (dei farabutti) è «in cima ai miei pensieri. L'attuale disegno di legge non risolve tutti i problemi, ma è un primo passo importante: cercheremo di migliorarlo più avanti». «Solo una piccola *lobby* di magistrati e giornalisti è contraria alla legge sulle intercettazioni. La grandissima maggioranza» (dei farabutti, dei ladri, dei corrotti e dei corruttori, degli omicidi, dei peculatori, dei falsificatori, e compagnia varia) «è stanca di non poter usare il telefono per tema di essere spiata» Oggi i malfattori stano canticchiando: «Meno male che Silvio c'è». È diventato il loro inno. Unitevi anche voi al coro, alla faccia degli italiani imbrogliati. Non so se i sacerdoti della fiducia siano collusi o pavidi; sono certamente complici e conniventi. Vergogna! Non bisogna però rinunziare alla resistenza e alla lotta. Assisteremo al giorno in cui tutto il crepuscolare basso impero berlusconiano sarà inghiottito dall'ignominia e ricordato come una parentesi nefasta per l'Italia. La resistenza si compie anche con gesti significativi e simbolici, come l'occupazione dell'Aula da parte dei senatori dell'Italia dei Valori; che, nel momento in cui si è proceduto, penso correttamente, alla loro espulsione, la stampa non abbia potuto assistere alla ripresa di sovranità di quest'Aula. Comunque, io condivido la battaglia del mio partito, perché quel gesto era volto a sottolineare con forza il nostro no al malaffare, il nostro no alla alla fiducia al Governo protettore del malaffare, il nostro sì all'onestà, alla speranza, al lavoro, ai sacrifici del popolo italiano. Viva l'Italia onesta e pulita! Signor Presidente, colleghi senatori, siamo qui per confermare, nostro malgrado, il giudizio negativo sulla legge di riforma delle intercettazioni. Nostro malgrado, perché, com'é noto, sul tema della riforma della giustizia abbiamo sempre ritenuto che il Parlamento, maggioranza ed opposizioni insieme, debba fare un vero e proprio salto di qualità, evitando di trasformare le istituzioni rappresentative (come purtroppo anche questa volta è avvenuto e come puntualmente avviene ogni qual volta si discute di giustizia) in un'aula di tribunale nella quale si misurano solo i rapporti di forza tra i sostenitori della difesa ed i sostenitori dell'accusa. Noi non siamo iscritti né al sindacato dei magistrati né al sindacato degli avvocati e men che meno a quello degli imputati. Noi aspiriamo a rappresentare i cittadini, il popolo italiano, nel nome del quale si dovrebbe sempre e solo amministrare la tutela dei diritti. Purtroppo, questo Paese da tanti anni non riesce ad avere una seria riforma della giustizia, una riforma che vada nella direzione giusta e cioè nella direzione di garantire i diritti di libertà dei cittadini e tra questi, innanzitutto, il diritto alla sicurezza. Purtroppo, in questi anni, le modifiche alla legislazione sono avvenute solo per rendere ancor più vischioso il sistema giudiziario e più funzionale ora agli interessi della magistratura ora a quelli dell'avvocatura, mai per rendere più agevole al cittadino l'accesso alla tutela dei diritti e più efficiente la macchina giudiziaria che è la parte più complessa e delicata dell'amministrazione dello Stato. Anche la legge che ci proponete non sfugge a questa drammatica constatazione, perché ci state costringendo ad approvarla così com'è, ricorrendo al voto di fiducia. A tale riguardo, consentitemi di dire, senza polemica e senza la falsa indignazione di quanti amano indulgere alla piazza piuttosto che assumersi la responsabilità di decidere in Parlamento come migliorare le condizioni del Paese, che non ha senso né politico né istituzionale porre la fiducia qui in Senato sterilizzando il confronto parlamentare proprio nel momento in cui quest'ultimo poteva svoltare positivamente nel senso di una convergenza più ampia. La questione di fiducia posta così a freddo è solo un atto di forza che nasconde insicurezza e debolezza. La fiducia non era necessaria soprattutto dopo che la maggioranza (siete 100 più di noi) ha raggiunto l'intesa su di una proposta. Quest'ultima avreste dovuto offrirla al contributo delle opposizioni, senza chiudervi a riccio. Così facendo, cari colleghi, avete commesso due errori: avete mostrato che al vostro interno la coesione rischia di durare lo spazio di un mattino (e per questo vi state affrettando a licenziare un provvedimento costi quello che costi); costi); avete chiuso ogni dialogo con le opposizioni, anche con quelle più aperte al confronto e alla discussione, mettendo sullo stesso piano «sciacalli e leoni». A cosa vi serva tutto ciò sinceramente stentiamo a comprenderlo. Non serve, certo, a rendere più disteso il clima politico di un Paese chiamato a compiere proprio in questi giorni enormi sacrifici. Un Paese che ha bisogno dell'apporto di tutti per superare le difficoltà che si trova davanti. Non serve a rendere più agevole il dialogo tra le forze politiche, così come auspicato dal nostro Capo dello Stato, che con fatica si spende quotidianamente per rendere le istituzioni più credibili e più vicine ai bisogni della gente. Ci avete chiuso la porta in faccia proprio nel momento più propizio, in cui le vostre aperture al confronto avevano indotto, anche noi, a ritenere possibile la convergenza su un testo migliore ed ampiamente condiviso. Eppure noi abbiamo lavorato solo per migliorarlo questo provvedimento, perché riteniamo giusto tutelare i cittadini dall'abuso d'informazioni riservate, dall'uso strumentale della *privacy* a fini politici o di estorsione, dalla indebita intrusione nella loro vita senza che vi sia una buona ragione per farlo. Riteniamo, infatti, fondata un'iniziativa legislativa che sia animata da sinceri sentimenti di riequilibrio tra due interessi costituzionalmente protetti: la dignità della persona umana e la sicurezza pubblica. E, quindi, una nuova disciplina delle intercettazioni che, senza pregiudicare il diritto-dovere dei magistrati di investigare, intervenga sull'abuso di questo indispensabile mezzo di ricerca della prova ci sembra quanto mai opportuna. Ma una disciplina che limiti appunto l'abuso e non anche l'uso di questo indispensabile strumento d'indagine. Noi abbiamo viceversa un testo che, pur con cambiamenti e ripensamenti della maggioranza, è ancora squilibrato. Perché affidare a un tribunale collegiale l'autorizzazione ad intercettare anche per i reati più gravi significa rendere difficile al pubblico ministero il ricorso alle intercettazioni quando vi sono in ballo delitti gravi e di particolare allarme sociale; significa rendere più difficile la celebrazione dei processi per quei reati moltiplicando il numero dei giudici incompatibili, significa introdurre un sistema irragionevole in forza del quale basta un solo giudice a condannare all'ergastolo un cittadino e ce ne vogliono tre per fare le intercettazioni che servono a portarlo in giudizio da quel singolo giudice; significa trasformare l'intercettazione da mero strumento di ricerca della prova a prova regina differenziando il regime giuridico che riguarda questo strumento dagli altri strumenti di ricerca della prova parimenti intrusivi della *privacy* come l'ispezione, il sequestro, la perquisizione. Ma, cari colleghi della maggioranza, vi sembra meno intrusiva un'ispezione personale, con tanto di verbale piazzato sui giornali, che svela pregi e difetti fisici della persona ispezionata? Noi crediamo di no e, quindi, ci appare irragionevole una disciplina differenziata per eguali mezzi di ricerca della verità. Ed ancora, vi sembra giusto l'aver equiparato alle intercettazioni telefoniche le intercettazioni ambientali, l'acquisizione dei tabulati telefonici e le videoriprese? Questi ultimi sono strumenti certamente meno invasivi della *privacy* e viceversa assolutamente indispensabili nella lotta alla mafia e al terrorismo. Questo vostro modo di disciplinarli rende difficile e a volte impossibile a forze dell'ordine e magistratura perseguire tali reati con efficacia e tempestività. E che dire del limite rigido di durata delle intercettazioni? Siete stati costretti, e ve ne diamo atto volentieri, a rivedere questa norma dalle conseguenze allucinanti. Se, infatti, al settantacinquesimo giorno di ascolto di un pregiudicato si scopre che il giorno successivo commetterà un omicidio, non si sarà in condizioni di arrestarlo perché non si possono più ascoltare le sue conversazioni. Ma il rimedio che avete introdotto è peggiore del male perché costringete il pubblico ministero a dover adottare ogni 72 ore provvedimenti urgenti che un tribunale collegiale dovrà in tempo reale convalidare. Mi chiedo e vi chiedo: e se nei tre giorni d'intercettazione disposta con urgenza dal pubblico ministero non interviene la convalida del tribunale (per il carico di lavoro, per i tempi di trasmissione o di esame della documentazione o per altre ragioni obiettive che ne impediscano la decisione in tempi così stretti) cosa succede? Si brucia così, per un disguido burocratico, un'indagine delicata? E cosa raccontiamo alle vittime di reato? Che per mancanza di un'auto di servizio, di una fotocopiatrice o per l'indisposizione di un magistrato le intercettazioni che sono servite ad arrestare il loro aguzzino non possono essere usate per condannarlo perché un tribunale le ha autorizzate fuori tempo massimo? Su questo aspetto potevano fare di più e di meglio se solo ci aveste messo nelle condizioni di discuterne insieme. Che senso ha, cari colleghi, precludere alla libera stampa l'accesso alle aule di un tribunale per raccontare l'udienza di un processo che tanto scalpore ha suscitato nell'opinione pubblica? A quale logica obbedisce tutto ciò, visto che proprio perché il dibattimento è pubblico ampia deve essere la sua diffusione per un principio di trasparenza dell'azione della magistratura e di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, che appunto si amministra nel nome del popolo italiano? E perché consentire, a causa di un mero atto dovuto qual è l'iscrizione nel registro degli indagati, la sostituzione del pubblico ministero che ha condotto le indagini se non per sbarazzarsi di un giudice scomodo che conosce le carte dell'indagine e che quindi può sostenere con vigore le tesi accusatorie nel processo? A queste domande non è stato possibile dare una risposta compiuta perché avete posto la fiducia impedendoci di migliorare il testo del disegno di legge. Anche sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni si poteva e si può migliorare il testo. Se, infatti, in un primo momento le sanzioni nei confronti della stampa sono state ridimensionate, non si capisce perché da ultimo avete introdotto, senza alcuna possibilità di discuterne, un emendamento che introduce ulteriori sanzioni penali nei confronti degli editori. Vi rendete conto che così incidete profondamente nell'assetto proprietario delle aziende editoriali e nel delicato rapporto tra editore e giornalista? Vi abbiamo proposto tante soluzioni, anche molto equilibrate, a cui non avete potuto (e forse non avete voluto) dare ascolto. ascolto. Signor Presidente, credo che anche sulle spese delle intercettazioni si poteva fare di più. Noi siamo convinti che su questo fronte vi sono stati evidenti eccessi e ciò perché vi sono, come ha detto il ministro Alfano, 2.000 centri di spesa che non hanno parametri oggettivi e predeterminati per valutare la congruità

le indagini. Signor Presidente e cari colleghi, eravamo pronti a discutere senza riserve in quest'Aula il testo concordato dalla maggioranza, che contiene alcuni importanti ed apprezzabili elementi di novità, e siamo rimasti basiti per il fatto che improvvidamente avete posto la fiducia. Non siamo indignati anche perché non siamo ipocriti; siamo meravigliati per questo improvviso gesto di chiusura. Non intendiamo però rassegnarci e quindi alla Camera riproporremo le nostre proposte di modifica con lo stesso spirito costruttivo. Oggi votiamo contro, ma se alla Camera la maggioranza accoglierà i nostri emendamenti siamo pronti a cambiare

Primo: il testo della legge risponde alle esigenze delle forze di polizia che utilizzano le intercettazioni come strumento di indagine e allo stesso tempo però va a tutelare la *privacy* dei cittadini limitandone gli abusi del passato. Secondo: con questo voto andremo anche a stoppare le tante, troppe e in molti casi strumentali polemiche sollevate dalla discussione di questo disegno di legge. I cittadini sono stanchi, stufi, non ne possono più di assistere a continue liti, a contrasti inutili nelle Aule parlamentari, che alla fine fanno perdere solo tempo. *(Applausi è da due anni che discutiamo in Parlamento di intercettazioni: troppo tempo! Con il voto di oggi il Senato potrà finalmente dedicarsi ad altro, *in primis* alla manovra fiscale, provvedimento che noi consideriamo invece necessario ed urgente per contrastare la crisi economica che stiamo vivendo e rilanciare la crescita del nostro Paese. Le opposizioni si sono inventate di tutto per allungare i tempi di discussione di questo provvedimento sulle intercettazioni allo scopo di affossare questa legge. Un atteggiamento legittimo, che noi però consideriamo sbagliato, proprio di chi non sa far altro che cavalcare il dissenso. Ma definirla una legge che favorisce le mafie, colleghi del centrosinistra, è davvero troppo. In queste parole c'è tutta la vostra malafede. *(Commenti dal Gruppo PD).* E per dimostrare che le vostre sono solo bugie e falsità, basta guardare ai fatti. Questo, cari colleghi, è il Governo che ha portato a casa i risultati migliori in tema di contrasto alla criminalità rispetto a tutti i Governi che lo hanno preceduto. I fatti parlano chiaro: centinaia e centinaia di latitanti arrestati, intere cosche sradicate, miliardi di euro in beni sequestrati alle mafie. Ma non solo: con l'introduzione del pacchetto sicurezza voluto dal ministro Maroni abbiamo bloccato i flussi di clandestini in arrivo sulle nostre coste; i reati sono diminuiti e le nostre città oggi sono più sicure. Questa è la realtà. Anziché accusare noi di aver fatto una legge che favorisce le mafie, pensate a quello che avete fatto voi con il Governo Prodi. Con il vostro Governo, cari colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, avete fatto aumentare la criminalità in maniera esponenziale. Basta ricordare gli sbarchi quotidiani a Lampedusa di carrette del mare stracolme di extracomunitari clandestini, che poi da lì si trasferivano direttamente nelle nostre città, dove vivevano nell'illegalità e in molti casi delinquendo, dedicandosi allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione, ai furti negli appartamenti, alle rapine. *(Commenti del senatore Maritati).* Non contenti di questo, avete voluto e votato l'indulto (ricordiamocelo), scarcerando così migliaia e migliaia di delinquenti che hanno ricominciato a commettere reati. Con il vostro Governo, cari colleghi dell'opposizione, non siete stati in grado di arrestare i latitanti, che noi abbiamo arrestato, e di sequestrare i patrimoni illeciti dei mafiosi, che questo Governo ha sequestrato!

I mafiosi stavano meglio quando c'eravate voi al Governo. Questa è la realtà

Prego, senatore Bricolo, continui. BRICOLO *(LNP)*. Ma come me la pensano i milioni e milioni di cittadini di questo Paese che, con il loro voto, anche per questi motivi, hanno deciso di non farvi più governare. Siete all'opposizione perché l'hanno deciso i cittadini: ricordatevelo!

anni fa fu lo stesso Indro Montanelli a denunciare, per primo, il vergognoso abuso che i giornali facevano delle intercettazioni. Aveva ragione, ed ora la situazione è sicuramente peggiorata. Siamo di fronte ad un *Far West* dove tutti possono essere intercettati, anche senza motivo. Il nostro Paese ha il record per quanto riguarda le utenze intercettate, che sono molte di più di quelle di Francia, Germania e Inghilterra messe assieme, e cinquanta volte di più che negli interi Stati Uniti d'America. Visti i numeri esorbitanti, ovviamente la stragrande maggioranza di queste intercettazioni è inutile, però costa. Il Ministero della giustizia ha un debito di 500 milioni di euro, mille miliardi di vecchie lire, da pagare alle ditte che le fanno su richiesta delle procure. Per di più, si doveva interrompere - a nostro avviso - lo scandalo di quei magistrati che, in palese violazione del segreto, girano ai giornalisti amici stralci di intercettazioni che magari non hanno alcun rilievo penale, semplicemente per screditare qualcuno, il loro nemico di turno. Troppi abusi e troppe irregolarità, che hanno messo a repentaglio la *privacy* dei cittadini, soprattutto di quelli estranei alle vicende giudiziarie. Allo stesso tempo, però, dovevamo garantire l'uso delle intercettazioni per le indagini, strumento che consideriamo indispensabile perché efficace, funzionale ed utile per la ricerca delle prove. Non è stato facile, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare ad un testo che consideriamo equilibrato, che va a bilanciare l'esigenza di assicurare l'efficienza delle indagini e l'esigenza di tutelare le garanzie individuali. E allora è giusto Tutti i reati che potevano essere finora intercettati rimarranno intercettabili: tutti, con l'aggiunta dello *stalking*, che non era previsto. Per quanto riguarda mafia, terrorismo e i reati di più grave allarme sociale, nessun limite alle intercettazioni. giorni più proroghe motivate all'infinito per gli altri reati, come avviene già in tutti i Paesi europei. Le intercettazioni ambientali si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di reato. Le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate per provare anche un altro reato. Le riprese video ed audio dei processi continueranno ad essere garantite. Per quanto riguarda i processi in corso, le intercettazioni già effettuate saranno tutte salve. Per intercettare una persona non si richiederà una prova di colpevolezza, nemmeno indiziaria, ma solo un vaglio serio delle esigenze investigative. Nulla di scandaloso, dunque, come affermano invece i colleghi dell'opposizione. Nessun aiuto alle mafie, anzi, finalmente norme chiare che regolano l'attività di indagine, con l'aggiunta ‑ è giusto ricordare anche questo ‑ di nuove regole per la pubblicazione sui giornali, con lo scopo di garantire il doveroso diritto di cronaca, evitando però gli errori del passato. Sono previste multe agli editori che pubblicheranno intercettazioni di cui è stata ordinata dai magistrati la distruzione. Infine, è giusto ricordare anche che tutte queste norme sono state introdotte qui al Senato, migliorando di gran lunga il testo già approvato dalla Camera, a dimostrazione che la maggioranza ha non solo ascoltato ma anche recepito le richieste che venivano dal Paese, dai Gruppi parlamentari, anche da quelli delle opposizioni, dalle forze di polizia, dagli editori, allo scopo di migliorare il provvedimento. Voglio dunque ringraziare tutti i Senatori della Commissione giustizia per il lavoro fatto e anche chi ha sempre cercato la giusta mediazione fra maggioranza e opposizione allo scopo di evitare il più possibile inutili scontri e contrapposizioni: il presidente Schifani. Con l'approvazione di questo provvedimento, come ricordavo precedentemente, finiranno finalmente anche le polemiche e gli scontri d'Aula sulle intercettazioni e potremo passare finalmente ad altro. La fiducia si è resa necessaria anche per questo. Potevamo perdere altre settimane di tempo votando in Aula centinaia e centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni, ma dopo due anni di contrapposizione muro contro muro, francamente si rischiava solo il blocco dell'attività parlamentare: e questo, cari colleghi, non possiamo permettercelo. Il Paese non può permetterselo. Finalmente potremo dedicare il nostro tempo a discutere della manovra fiscale. Su questo chiediamo il contributo di tutti, anche delle opposizioni. Non serve protestare solo in piazza. Chi ha idee e chi ha proposte costruttive le può presentare in Aula, e insieme siamo disposti a condividerle.

il Paese aveva bisogno di una riforma delle intercettazioni telefoniche. Ne aveva bisogno perché è intollerabile che sulle pagine dei giornali appaiano notizie che o sono coperte dal segreto istruttorio

È intollerabile che si faccia mercato della dignità dei soggetti ed è intollerabile che vi siano fughe di notizie rispetto ad atti investigativi che probabilmente vengono frustrati nella loro efficacia dalla fuga di notizie stesse. Aveva davvero bisogno una buona legge, tanto è vero che già dai primi atti del governo Prodi della scorsa legislatura, con un disegno di legge Mastella e poi, di nuovo, in questa legislatura, con due proposte di legge, una delle quali firmata dalla Capogruppo, noi abbiamo chiesto la riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche. Cosa dovevamo fare? Cosa pensavamo che dovesse fare una buona legge sulle intercettazioni telefoniche? Innanzitutto, consentire la pubblicazione delle intercettazioni, ma solo se esse sono pubbliche (cioè già a conoscenza dell'imputato e del suo difensore) e se sono quelle già selezionate dal giudice, che avrebbe dovuto selezionare tutte quelle (per legge, naturalmente, con delle sanzioni, se non lo faceva) che erano o non pertinenti al processo lesive, rispetto alle indagini, della dignità, della *privacy* dei soggetti o addirittura riguardanti soggetti del tutto estranei alle indagini. Bisognava consentire la pubblicazione degli atti, ma solo di quelli non più coperti da segreto, naturalmente, perché questa è ancora una questione equivoca - come sanno i colleghi della maggioranza - sulla quale la giurisprudenza ha qualche incertezza ed era bene scriverlo nero su bianco.

eliminato da quelle che potevano essere utilizzate. Quindi, una buona legge sulle intercettazioni telefoniche che tutelasse la *privacy* e la dignità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle indagini.

Innanzitutto, perché questa legge limita l'uso delle intercettazioni telefoniche come strumento di acquisizione della prova. Lo limita per i presupposti che prevede; lo limita nella durata; lo limita individuando un giudice competente che sta nell'ufficio del distretto (e quindi con una fuga di notizie, visto che questi faldoni viaggeranno da una città all'altra e continuamente); lo limita perché solleva il giudice che abbia detto «Io sono il giudice di questo procedimento»; e, con la nozione vaga che avete inserito nella legge, ovviamente lo limita per ogni questione. Lo limita perché limita, e gravemente, per esempio, la possibilità di ricorso alle intercettazioni ambientali, che oggi sono permesse solo per tre giorni e soltanto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per i reati comuni. Ricordate il caso di Novi Ligure? La chiacchierata tra Omar ed Erika? Ecco, ora non sarebbe più captabile, così come non sarebbe captabile ciò che si dicono due pregiudicati nella cella di un carcere. E poi bisogna comunque avere, anche per questi tre giorni e questa miserrima intercettazione ambientale, una prova diabolica: il giudice deve prevedere che ci saranno elementi fondamentali per l'accertamento del reato o deve impedire la commissione del reato. Avete equiparato intercettazioni, videoriprese non captative - parola complicata, che capite da soli - e anche tabulati, anche se la Corte costituzionale aveva detto che per i tabulati tutta questa esigenza di *privacy* non c'era. Potrei continuare, ma c'è un secondo punto. Questa è la vostra legge, guardate: punite la pubblicazione di atti di indagine e consentite solo la pubblicazione per riassunto fino alla fine delle indagini preliminari. Ma vi rendete conto dell'arbitrio che il giornalista può compiere per riassunto? Non voglio irritarvi, ma il caso Boffo e «il Giornale» lo ricordate o no? Ed impedite anche la pubblicazione, fino alla fine delle indagini preliminari e salvo per riassunto, anche degli atti che non sono segreti, che sono pertinenti alle indagini e che non sono lesivi della dignità e onorabilità dei soggetti. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, non si può pubblicare assolutamente alcunché. Punite anche gli editori, perché casomai il giornalista o il direttore del giornale largheggiasse nell'informazione pubblica - ohibò! - interviene l'editore del giornale e dice: ma che, mi volete far fallire? E di conseguenza, l'editore

Concludendo, questo tutela meglio la *privacy* dei soggetti? No. Questo tutela meglio, molto meglio, i criminali. Questo uccide il diritto dei cittadini ad essere informati. Questo provvedimento uccide la libertà di informazione tutelata dalla Costituzione. una sola volta, presidente Berlusconi, perché mentre la parola «impresa», in varie forme, appare almeno tre volte nella Costituzione, le parole «libertà personale» e «libertà d'informazione» esistono una sola volta perché chi si sente vincolato alla Costituzione lo sa che non c'è bisogno di ripetere ciò che è sacro! È una commedia degli equivoci plautina la vostra, colleghi. E allora, senatori del PdL, chi oggi vota la fiducia, vota la limitazione della libertà di informare e di essere informato, la limitazione dei mezzi a disposizione degli investigatori per accertare reati, per individuare i colpevoli, per punirli. E il presidente Gasparri e il vice presidente Quagliariello la finiscano con la storia delle intercettazioni negli Stati Uniti: è una balla! Dall'inizio della crisi economica è aumentato del 26 per cento il numero delle intercettazioni disposte con una equiparazione dei mezzi di intercettazione intercettazione a disposizione degli investigatori per accertare i reati finanziari, che risultano identici a quelli adoperati per tutelare la sicurezza nazionale e contrastare il crimine organizzato. E i numeri che danno sono sballati per una ragione semplice: che viene data una sola autorizzazione per intercettare tutti gli imputati, una media di 113 per processo, e che l'autorizzazione a intercettare non ha limiti di durata e comprende tutte le possibili forme di intercettazione. Quindi cercatevi un altro paragone, perché questo non funziona. La verità allora è davvero un'altra: voi avete colto l'occasione, in un momento assai imbarazzante, diciamo così, per il Governo e per la maggioranza, di nascondere agli italiani i pubblici misfatti, l'esercizio deviato dei pubblici poteri, l'uso privato e la dissipazione delle pubbliche risorse. Voi volete nascondere, voi vi nascondete. Voi non volete controllo (ma questo lo sapevamo già): il popolo che citate così spesso lo volete cieco e sordo, manipolabile. Voi vi servite del popolo quando vi serve per celebrarvi, ma lo volete bue. La *privacy* che dite di tutelare è la vostra, è l'ombra nella quale volete continuare a fare i vostri affari. Chi si accontenta nella maggioranza, chi fa finta di non saperlo, oggi non può non saperlo. Io che tremo - non come voi, che l'adoperate in maniera sguaiata e volgare - quando pronuncio la parola libertà, non in nome mio ma in nome d'altri, vi dico che qui il mio Gruppo, che mi ha dato mandato sulla base di un'assemblea che abbiamo celebrato, non parteciperà al voto di fiducia. Non parteciperemo perché noi vogliamo che risulti con ogni evidenza e con il rispetto sacro che abbiamo di quest'Aula e della legge il fatto che da qui comincia il massacro della libertà.

Ma noi parliamo, oltre che al Parlamento e al Governo, al Paese. Qualche attimo fa voglio darne atto, il senatore Li Gotti, ha riscontrato la correttezza delle procedure. Alcuni colleghi dell'Italia dei Valori avevano occupato l'Aula ed occupato i banchi del Governo; si è dovuto differire di qualche minuto l'inizio del voto per poter sgomberare l'Aula. Siccome fuori dall'Aula qualcuno protesta, si è dato atto da parte di quel Gruppo in quest'Aula della correttezza delle procedure. Il Parlamento si rispetta con la presenza, con il voto e con il dibattito.

Noi siamo orgogliosi delle modifiche che abbiamo apportato anche con la discussione con la società civile, con le realtà del mondo delle professioni e financo all'interno della maggioranza, all'interno di un grande partito: il Popolo della Libertà è il primo partito d'Italia perché sa confrontarsi e sa applicare al suo interno il metodo della democrazia che voi oggi ancora una volta ignorate e calpestate.

abbiamo registrato tante dichiarazioni importanti. Un uomo della sinistra come Giuliano Pisapia ha detto che una legge come questa era necessaria,

la Corte costituzionale, con una sentenza sul diritto di cronaca, aveva detto che era legittimo il divieto di pubblicare atti processuali fino al termine delle indagini, proprio perché le pubblicazioni favoriscono i criminali. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Quindi è pubblicare tutto che aiuta il crimine e non mettere delle regole alle pubblicazioni. Noi attuiamo, forse in ritardo, una sentenza della Corte costituzionale del 1995. Per quanto riguarda i dati che sono stati citati, sappiamo che l'Italia è il Paese di mafia, camorra e 'ndrangheta e quindi il numero delle intercettazioni, a volte, cresce a causa di questi fenomeni criminali.

ogni 100.000 abitanti. Anche negli Stati Uniti confermiamo che il numero delle intercettazioni è largamente inferiore a quello dell'Italia e negli Stati Uniti e altrove l'intercettazione è *l'extrema ratio* dell'attività investigativa, non c'è l'uso strumentale e costante, l'abuso dell'intercettazione che si fa in Italia. Gherardo Colombo, un ex magistrato, giorni fa ha detto: Si usino di più altri mezzi, è più faticoso, ma è importante farlo. Non sempre e non solo l'intercettazione. Sull'informazione, un maestro di giornalismo come Piero Ostellino ha scritto il 23 maggio, sul «Corriere della Sera», che: «I processi, in uno Stato di diritto, si fanno in tribunale e non sui giornali, alcuni dei quali inclini per ragioni editoriali o politiche a fare strame

quando ha detto che una legge era necessaria, perché non c'è la capacità del mondo delle professioni di autoregolamentarsi. «Abbiamo pubblicato intercettazioni inutili, coinvolgendo persone estranee alle indagini per storie pruriginose»: lo ha ammesso

domiciliari a Bari, il quale in una telefonata con una giornalista riferisce alcune notizie di interrogatori e poi le passa il magistrato, che dice alla giornalista: «Tutto bene? Come sarà l'articolo?». Io sono un giornalista professionista: giornalisti che lavorano in questo modo sono la vergogna del giornalismo italiano. Questo non è giornalismo. L'inchiesta che è in corso a Trani riguarda anche Trani riguarda anche un magistrato: lo si legge sui giornali. E sapete chi era l'obiettivo? Indovinate un po'? Silvio Berlusconi, che non ha commesso nessun reato, ma bisogna usare intercettazioni, rapporti e contiguità

«Altro che multe da 3.000 e 5.000 euro: noi li dobbiamo chiudere quei giornali» disse D'Alema. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Ecco, io dico a D'Alema che noi difendiamo quella libertà di stampa che dà fastidio a lui e alla sua cultura politica. Ci riveli lui qualche segreto italiano su tante vicende che attendono ancora una parola una parola di verità, dal fondo Oak a tanti altri fatti su cui la stampa poco scrive in questo Paese.

sarebbe finita la lotta alla mafia, ma non è stato così. Vi arrabbiate perché rivendichiamo il numero degli arresti dei mafiosi (otto mafiosi al giorno, da quando siamo al Governo, ha fatto bene il presidente Bricolo a ricordarlo, miliardi e miliardi di

confronti dei latitanti, non ci sono limiti, nulla è stato modificato, si può intercettare e indagare *ad libitum*, per garantire la sicurezza dello Stato.

le intercettazioni a strascico. Abbiamo introdotto meccanismi più attenti e severi. Non ci sarà peraltro la sostituzione automatica del PM: ciò dimostra che abbiamo ascoltato le osservazioni ragionevoli, quando sono state formulate. Abbiamo voluto ricordare che, nella Costituzione repubblicana, oltre all'articolo 21 - sacrosanto - sulla libertà di espressione, c'è anche l'articolo 15, il cui testo voglio leggere a conclusione del mio intervento: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Vogliamo coniugare la libertà dell'investigazione e la persecuzione dei reati con la libertà del cittadino. Siamo quindi nel solco della Costituzione, nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale e pertanto votiamo sì, orgogliosi e convinti come sempre, su questa legge!

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi senatori radicali parteciperemo alla votazione e voteremo convintamente no. A volte, presidente Gasparri, alzare la voce e urlare serve a coprire l'inconsistenza e la fragilità delle motivazioni. Colleghi, per cortesia. BONINO *(PD)*. No. Il decoro e l'attenzione istituzionale che abbiamo sempre dimostrato li potreste anche guardare con un po' più di rispetto. Scusatemi, colleghi! Voteremo no perché non abbiamo fiducia nel merito delle politiche che di volta in volta proponete, anzi imponete, a questa Assemblea, a cominciare da questa. Ma di quale tutela della *privacy* parliamo, senatore Gasparri? Cosa c'entra? Avete tolto persino la registrazione audio di Radio Radicale dei processi. Che cosa c'entra questo con la *privacy?*

perché, signori del Governo, signori colleghi, non è possibile sentire da voi - e da molti, tra l'altro come «libertà d'informazione», «libertà e correttezza dell'informazione», che questo Paese non sa neppure cosa siano da tanto tempo, tra lottizzazioni, occupazioni, usurpazioni di tutti gli spazi possibili e relative espulsioni di tutti coloro che, non conniventi e neppure complici, esprimono idee diverse. Ma un no, presidente Gasparri e Governo, ancora più convinto è al metodo, che è fuori da qualunque accettabile procedura regolamentare con cui governate, con cui avete governato questo procedimento in una china rovinosa in cui trascinate anche le istituzioni parlamentari. Per questo motivo, esprimiamo il

anzi, in un sistema democratico i diritti inalienabili non si mettono mai neppure ai voti. Ci sono invece diritti costituzionali che in questo provvedimento avete negato e calpestato. Per questo, il nostro no, rispettoso delle istituzioni, è decisamente convinto nel merito.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È estratto

Alberti Casellati, Alicata, Allegrini,

dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.